La seduta è ripresa. Onorevoli colleghi, comunico che, come già preannunciato ieri alla Conferenza dei Capigruppo, all'inizio della seduta pomeridiana di domani, giovedì 16 novembre,

il Ministro della giustizia, richiesto sia in Commissione che in Aula, in occasione della discussione su tale provvedimento, dei dati relativi alla stima degli scarcerati a seguito dell'indulto, fornì una cifra che si aggirava attorno alle 12.000 unità e i verbali lo confermeranno. Dai banchi di Alleanza Nazionale già allora si mossero delle riserve sul punto, proiettando invece questa stima alle 24.000 unità. Da tempo il numero indicato dal Ministro della giustizia è stato superato. Ieri, abbiamo assistito a un confuso alternarsi di numeri: 17.000, 29.000, 24.000 a seconda di quale fosse la fonte. Non entro ovviamente nel merito della stima (non è questo il momento), però ritengo sia indispensabile che, su una questione così delicata, ci sia una parola chiara da parte del Governo. Non credo sia vietato discutere e avere notizie su questa materia per il solo fatto d'indulto è stato approvato da più dei due terzi dei parlamentari, perché è ovvio che, se quello era il *quorum*, si dovessero superare i due terzi. Ritengo, anzi, che tutti siano legittimati ad avere questa chiarezza di dati, anche coloro che hanno votato a favore dell'indulto (io non era tra questi), perché il loro voto può essersi formato anche sulla base della stima fornita dal Ministro della giustizia. Allora, poiché quei dati sono certamente falsi (quelli del 29 luglio), poiché il Ministro dell'interno è venuto a raccontarci soltanto le sue sofferenze, credo che solo il rigore del Presidente del Consiglio - che è particolarmente versato nel dare numeri, soprattutto in questo periodo - possa risolvere la questione.

Vorrei associarmi alla sua richiesta, perché qui ci troviamo di fronte ad un caso che credo sia ancora più grave. Per quale motivo? caso unico, o sicuramente raro, nel panorama ministeriale italiano, tutta la rete dei penitenziari del nostro Paese è collegata in via informatica in tempo reale. significa che, se vi è un dato in tutto il Ministero della giustizia assolutamente preciso e aggiornato, minuto per minuto, è proprio quello sull'uscita e sull'entrata dei detenuti. Ogni ora, il dato preciso di quanti detenuti permangono all'interno dei penitenziari italiani, di quanti ne sono entrati e di quanti ne sono usciti. La sensazione di questo balletto di cifre,

avevamo previsto esattamente che il numero di detenuti che sarebbero usciti sarebbe stato molto, ma molto superiore ai 12.000 che il sottosegretario Manconi aveva

degli effetti del provvedimento di clemenza adottato nello scorso luglio sia il Ministro della giustizia. peraltro, che egli, già nel pomeriggio di ieri, ha fornito dati più puntuali ed esaurienti rispetto a quelli che, in modo intempestivo, confuso, contraddittorio ed improvvido, erano stati resi noti nella mattinata e nel primo pomeriggio In Commissione giustizia abbiamo fatto presente al Sottosegretario che rappresentava il Governo come quei dati fossero del tutto campati in aria. Egli ne ha preso atto, impegnandosi a fornirne più corrispondenti al vero. Perché i dati improvvidamente resi pubblici - non so bene se dal DAP o da uno dei Sottosegretari sono completamente campati in aria? Perché non era quello il numero delle persone effettivamente uscite dalle carceri italiane per effetto dell'indulto: nel calcolo di quelle cifre così alte erano state comprese persone persone già da tempo in circolazione, che non sono uscite dalle carceri per effetto dell'indulto. Ben venga un chiarimento ulteriore, non vedo l'urgenza sottolineata dal collega Mantovano: basta saper leggere le cifre e i dati forniti già ieri sera dal Ministro della giustizia. Voglio sottolineare come sia il caso di evitare, in futuro, che dati alla rinfusa, contraddittori e sbagliati, vengano resi noti da fonti che, comunque, sono ufficiali.

tenuto a riferire qui in Aula, e non solo sui dati definitivi per quanto riguarda le scarcerazioni dovute all'indulto, perché fino ad ora abbiamo dati confusi. Un Sottosegretario in Commissione giustizia ha fornito delle cifre completamente diverse da quelle che poi sono pervenute nel tardo pomeriggio di ieri dal Ministero della giustizia; ciò sta a significare lo stato di vera e propria confusione che regna in quel Ministero. signor Presidente, probabilmente se il Governo avesse fornito dei dati definitivi e completi sui livelli di scarcerazione all'interno del sistema della giustizia penitenziaria italiana, probabilmente l'indulto non ci sarebbe stato, perché si tratta di 30.000 scarcerati nell'arco di un anno. Quindi, anche le politiche di allarmismo sociale sulla tenuta del sistema carcerario

è detentrice di pacchetti di voti non indifferenti. Pertanto, l'indulto è stato un prezzo pagato a quell'accordo pre-elettorale che si è verificato in alcune aree del Sud.

di alcune zone (per esempio, per quanto riguarda la Puglia, quelli della provincia di Foggia) per capire che questo accordo, questa intesa, questo voto di scambio collettivo e di massa è stato anche il presupposto per il successo elettorale della sinistra nelle elezioni regionali pugliesi del 2005.

e ne spiego le ragioni. Su questo argomento credo dobbiamo stare molto attenti a non raccogliere informazioni non esatte e controllate e a non mettere in circolo una serie di apprezzamenti che disorientano la pubblica opinione. Noi siamo partiti, alcuni anni fa, da una dichiarazione del Ministero della giustizia, ripetuta sotto diversi Guardasigilli,

Noi avevamo una tradizione che risale alla monarchia e che la Repubblica ha conservato perché questi istituti ed il rispetto del precedente non cambiano con i mutamenti istituzionali. Ad un certo momento, però, abbiamo introdotto una garanzia, quella di richiedere una fortissima maggioranza parlamentare per poter dar vita a questo tipo di provvedimenti: questa - ripeto - è una garanzia.

non ho alcuna autorità per farlo, ma, siccome quello che noi diciamo ha una risonanza non solo nell'opinione pubblica, che si lascia un po' po' commuovere, qualche volta in bene, qualche altra volta in male, ma anche all'interno delle prigioni, noi dobbiamo avere un grande rispetto per gli uomini:

ringrazio, signor Presidente.

Signor Presidente, mi sembra strano un Parlamento che, dopo avere approvato l'indulto con una maggioranza dei due terzi, oggi si pianga addosso. Abbiamo avuto delle cifre drogate.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro della giustizia, l'UDC ha votato convintamente il provvedimento di indulto, anzi, avremmo, a suo tempo, votato anche un provvedimento più ampio che comprendesse l'amnistia. Devo dirle però oggi che lei, signor Ministro, ha una pessima strategia comunicativa oppure ha nel suo Ministero qualcuno che diffonde notizie contro la sua politica oppure - e forse è l'ipotesi più probabile - questo provvedimento di indulto è stato congegnato ed eseguito nel peggiore dei modi possibili. Infatti,

L'indulto senza amnistia ha provocato un intasamento degli uffici giudiziari, ma è impossibile, nello stato attuale della pubblica opinione, intervenire con un ulteriore provvedimento di amnistia, che verrebbe letto da tutti come una resa da parte dello Stato una resa da parte dello Stato davanti alla criminalità. Non risulta, poi, che siano state adottate misure adeguate per accompagnare chi usciva dalle carceri in modo da una sorveglianza adeguata per impedire che si commettessero nuovi crimini e per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, che è l'unica via attraverso la quale si esce dal mondo della criminalità. Per tutte queste ragioni, un provvedimento di clemenza, anche da noi approvato, si sta trasformando in un *boomerang* contro princìpi di civiltà giuridica, perché il Paese - se lei non se ne è accorto, signor Ministro, glielo dico io - è furibondo perché ha avuto l'impressione che siano stati rimessi per strada criminali senza alcuna garanzia adeguata per la protezione dei cittadini onesti. Aggiungo che è stucchevole il continuo ripetere che l'indulto era necessario per svuotare le carceri. Un Paese civile crea un sistema carcerario in grado di alloggiare tutti i delinquenti che è bene che stiano in galera e, secondo le mie private valutazioni, in Italia ci sono 80.000 persone che dovrebbero stare in galera, mentre c'è posto nelle carceri al massimo per 55.000-56.000 persone. Predisponiamo un programma che consenta di alloggiare nelle patrie galere, in condizioni umane, tutti quelli che è bene che nelle patrie galere stiano. Infine, ho sentito parlare del governatore Cuffaro.

è uno dei vizi più gravi della politica italiana, che ha portato a conseguenze delle quali dovrebbero vergognarsi coloro che ne sono stati autori, compresi alcuni presenti in quest'Aula; e, infine, che, per quanto mi risulta, Cuffaro è indiziato di altro e ben minore reato, certamente non di complicità con la mafia.

ritenendo le richieste che sono state fatte dai colleghi in merito al bilancio degli effetti del provvedimento dell'indulto sostanzialmente giuste. giuste. L'indulto è stato approvato dal Parlamento, come i colleghi sanno, a larghissima maggioranza, tuttavia, da parte di coloro che lo hanno sostenuto e anche di coloro che non lo hanno sostenuto, viene l'esigenza di una complessiva valutazione degli effetti di questo provvedimento, che va ben oltre il semplice dato numerico in merito alle scarcerazioni. Ritengo, sulla base dei dati che conosco, che già nel tardo pomeriggio di ieri e ancora questa mattina ho avuto modo di sentire dai giornali radio, il Ministro ed il Governo abbiano chiarito l'errore che era stato commesso; tuttavia, nella discussione che qui abbiamo svolto - cito tra tutti l'intervento del senatore Andreotti - sono state sollevate delle questioni inerenti ad una valutazione più generale, non strettamente numerica degli effetti del provvedimento, in riferimento alle forti preoccupazioni relative alla condizione di pericolosità sociale, di allentamento della sicurezza in alcune parti del Paese, in relazione alla situazione interna alle carceri, in relazione - il tema è stato sollevato autorevolmente dal Consiglio superiore della magistratura - allo svolgimento dei processi in corso. In virtù di tutte queste valutazioni, tutte più o meno accentuatamente preoccupate, penso che non sarebbe giusto rinsecchire l'eventuale valutazione sugli effetti di questo provvedimento ad un semplice dato, di cui pure si deve tenere conto e che deve essere preciso, relativo al numero degli scarcerati nel corso di questi mesi per effetto della legge sull'indulto. Esattamente quella complessità e quella problematicità degli effetti del provvedimento, che sono state richiamate dai colleghi, mi inducono a considerare positiva l'iniziativa che è stata adesso annunciata da parte del senatore Bianco, ma io inviterei, naturalmente me ne faccio portatore verso il Governo,

in relazione a ciò che il Parlamento, ripeto, a grandissima maggioranza, ha fatto. Non so se questa proposta possa essere accolta dal Governo; se così fosse, aggiornerei questa eventuale prosecuzione della discussione alla prossima settimana, chiedendo appunto all'Esecutivo di operare in questo modo, tenendo presente che certamente ciò non è possibile questa settimana, anche perché, come ho comunicato poc'anzi, nel pomeriggio di domani sentiremo

intervengo semplicemente per dire a lei e ai colleghi che, per quanto mi riguarda, già ho corrisposto ad una iniziativa e quindi bisogna valutare se

e maturate convinzioni sanpaoline che si stanno manifestando. Io voglio ringraziare, scusate, quelli che hanno votato il provvedimento, come me; voglio ringraziare oggi l'onorevole Pecorella che, in una intervista di grande intelligenza e lucidità, conferma il giudizio positivo suo e del suo Gruppo politico

e, come tale, il Ministro della giustizia esegue la volontà del Parlamento. Che poi in questa volontà, non tirandomi indietro, ci sia stata anche la mia volontà concorsuale, come senatore della Repubblica, ritengo di avere detto il mio sì in quella circostanza e lo farei anche in questa analoga circostanza. Quindi, non ripiego, a differenza di altre libere valutazioni e di sofferenze maturate da parte di alcuni, e confermo il mio sì.

Governo. Il Governo verrà quindi a dare spiegazioni. Voglio dire al mio amico Buttiglione, un po' inutilmente sarcastico e lezioso in questa circostanza,

consentire che, come è stato detto, le due Commissioni avviino la verifica e la valutazione degli effetti del provvedimento dell'indulto in tutti i suoi molteplici aspetti che qui sono stati richiamati. Successivamente - ma la richiesta viene fatta immediatamente dalla Presidenza del Senato - sollecitare il Presidente del Consiglio, e ovviamente lo stesso Ministro, ad intervenire in Aula per una discussione in tale sede qualora, per esempio, le risultanze

questo tipo di lettura del Regolamento è stato largamente attuato dall'attuale maggioranza quando era opposizione. Qui non si tratta di ostruzionismo, signor Presidente;

dei risultati elettorali: 200.000 voti in meno sono sempre 200.000 voti in meno, ecco perché la sinistra in questa Camera è minoranza elettorale ma maggioranza parlamentare. Signor Presidente, in realtà, in quest'Aula, in queste ore di dibattito, si sta consumando, tra l'indifferenza e la inconsapevolezza della stragrande maggioranza dei colleghi di maggioranza e opposizione,

da un'ideologia di classe degradata al chavismo**,** cioè a quella sorta di sinistra sudamericana che in Venezuela discrimina antropologicamente le varie componenti della società.

nasce da una interpretazione della società che discrimina tra i buoni (gli eletti) e i cattivi (i dannati).

questo Paese, creando le precondizioni di un'antropologia totalitaria. Ecco allora che si discrimina il docente della scuola paritaria, si privilegia il docente della scuola pubblica, si ghettizza il docente della scuola paritaria. È un tipo di lettura della società riscontrabile in tutti i provvedimenti di questo Governo: nella finanziaria,

che provengono dalle scuole paritarie. Ecco, dunque, qual è il fondamento di questo provvedimento. Guardate che questo provvedimento riguarda la scuola. Senatore Di Lello le ricordo che il suo schieramento ha stravinto le elezioni in Calabria e in provincia di Reggio Calabria, le ha vinte in Campania, in Puglia, quindi se vogliamo affrontare questo discorso lo affronteremo in Commissione antimafia con documenti e dati di fatto elettorali. Credo che non le convenga, senatore Di Lello. In conclusione, signor Presidente, ecco perché parlo in dissenso

di maturità come commissari interni. Francamente la giustificazione che il ministro Fioroni in Aula ha addotto, cioè di presunto contrasto con l'articolo 97 della Costituzione, appare assolutamente risibile. Dico al ministro Fioroni: non ci prenda in giro! L'articolo 97 della Costituzione dice che agli impieghi della pubblica amministrazione si accede tramite concorso. È evidente che una commissione di concorso non è un impiego presso la pubblica amministrazione. Dunque facciamo chiarezza su questo aspetto: credo che votare questo emendamento impedisca un vizio di costituzionalità su una norma che certamente discrimina e pregiudica immotivatamente, per ragioni meramente di carattere ideologico, gli insegnanti delle scuole paritarie.

il senatore Novi. Visto che il senatore Novi ritiene che stia avvenendo una discriminazione nei confronti degli insegnanti delle scuole paritarie in quanto portatori di un voto a favore del centro-destra, mi permetto

sia in comportamenti, sia in dichiarazioni rivolte alle loro scolaresche - ne ho la prova certa - sia nell'espressione elettorale, a favore del Governo del centro-sinistra, a favore di Prodi, a favore di questa maggioranza parlamentare, che evidentemente non è più maggioranza del Paese. Quindi, mi preme rilevare che forse sarà opportuno che i rappresentanti degli insegnanti delle scuole paritarie e segnatamente delle scuole cattoliche prendano atto di questa ennesima discriminazione ai loro danni, che viene

credo di avere la facoltà di intervenire una volta sola, al di fuori dei compiti che mi sono consentiti come relatrice, relatrice, cioè della relazione e della replica, ma la discussione sugli emendamenti è insistita - e ne capisco certamente le ragioni su un tema che ritengo fondamentale per la considerazione comune che dobbiamo avere dei fondamenti della Repubblica:

e nella maturità di una storia pluridecennale di presenza di scuole non statali, il tema della parità scolastica, ponendo le condizioni effettive per il suo riconoscimento. Quella legge n. 62, insieme con la Costituzione, è la bussola che ha guidato il Governo e questa maggioranza nel tracciare la strada maestra anche per gli esami di Stato. Vorrei ricordare che la normativa sugli esami di Stato che il Parlamento è chiamato di volta in volta ad aggiornare, e in questo momento ad approvare per il prossimo futuro, riguarda appunto gli esami di Stato cui sono chiamati gli studenti italiani al termine del corso di studi di scuola secondaria superiore.

Mi riferisco alla possibilità che commissari esterni della scuola paritaria possano entrare nelle commissioni di esame della scuola statale, perché naturalmente i commissari esterni della scuola paritaria sono insegnanti della scuola statale. Perché

Credo perché trattandosi di esami di Stato la Repubblica accerta i risultati dal punto di vista dello Stato e, fatte salve tutte le condizioni di parità, non si vede perché una parte degli insegnanti delle scuole paritarie debba andare a certificare gli esami i risultati acquisiti dalle scuole statali. Mi rendo conto che in questo dibattito, non so se in maniera strumentale, posso pensare in maniera assai convinta,

è un rispetto delle regole dello Stato, ripeto per l'ennesima volta, fatte salve tutte le condizioni di parità per quanto riguarda ovviamente gli studenti e l'organizzazione del lavoro delle scuole paritarie (e appunto in questo momento la verifica da parte dello Stato rispetta l'organizzazione autonoma e libera delle scuole non statali). Non vorrei che avessimo la tentazione inconscia, non dichiarata,

di quel tema sacro, che neppure oso pronunciare, che è il tema di Dio, il tema *teo*. Voglio dirvi, cari colleghi, che qualcosa di strano è successo anche nel nostro Paese se per sostenere le posizioni politiche è necessario usare i valori religiosi. *(Applausi Respingo, in termini politici e culturali, questa chiamata delle scuole non statali ad una sorta di assimilazione alle posizioni che qui vengono dichiarate dall'opposizione. La respingo politicamente, ma vi dirò di più. Sono persuasa che le scuole paritarie, e segnatamente le scuole cattoliche, hanno ben compreso quale sia la loro missione nella cornice dello Stato e della Repubblica e non hanno, per essere legittimate e riconosciute, bisogno di alcuna difesa strumentale. Non usate ciò che non va usato.

Presidente, colleghi,

e ad altri esponenti della maggioranza, di ragionamenti che non riescono a convincere nessuno. Sono convinto, senatrice Soliani, che lei non è con la coscienza a posto, pur avendola a posto, dopo quello che ha

Senatore Strano, la pregherei, per un doveroso rispetto nei confronti di tutti i colleghi, di attenersi ai giudizi politici, che possono essere anche i più drastici e i più severi sul merito della legge e degli interventi che hanno svolto i colleghi, ma di astenersi da giudizi e valutazioni sui sentimenti di fede religiosa e di coscienza di ciascuno di noi.

- recuperato il senso di quanto ho affermato; d'altronde, viviamo in un momento nel quale è consentito a qualcuno di piantare spinelli nelle fioriere e in Parlamento, in cui lo Stato decide

nel senso che lei mi dirà: «Bravo, sei stato nel tema». Se non lo sarò, mi bacchetterà alla fine e non nel mezzo del mio intervento. PRESIDENTE. Senatore

che io dicevo alla senatrice che è stata costretta ad un intervento perché, con la coscienza a posto, non si sente evidentemente tutelata da una maggioranza che sta ancora una volta ribadendo i suoi pregiudizi contro la scuola privata, contro la scuola cattolica, con un'invasione dello Stato nella sfera del cittadino e nella sfera della libera interpretazione di ogni cittadino. *(Applausi

il Governo e la maggioranza hanno ribadito che bisogna annientare il pianeta della scuola privata. Dov'è questa parità di cui lei parla, questa reciprocità, se fino ad ora ha dovuto ammettere che viene negata in questa fattispecie? La reciprocità non può essere ad intermittenza, non può essere fatta a tempo su alcuni atti e non su tutti. Se reciprocità vi è, vi deve essere anche negli esami di Stato. Non si capisce per quale motivo nella sfera privata debba intervenire lo Stato mentre nello Stato non possa intervenire, nel momento del giudizio, anche la sfera privata che, in parità e reciprocità, partecipa al pianeta scuola. La verità, mi avvio alla conclusione Presidente e la ringrazio per avermi dato la parola, è che, ancora una volta, vi è un disegno mirato della maggioranza e del Governo, iniziato oggi, contro la sfera della scuola privata e cattolica. Dico questo senza voler offendere la sua né la sensibilità di altri cattolici che all'interno della maggioranza e del Governo fanno il proprio dovere.

Senatore Malan, non mi risultava, dagli appunti che ho davanti a me, che fosse intervenuto su questo emendamento alcun senatore o senatrice del gruppo dell'Ulivo. Pertanto, ho considerato l'intervento della senatrice Soliani a nome del Gruppo dell'Ulivo. Lo abbiamo inteso come tale e infatti mi ripromettevo, qualora l'avessero chiesta, di non dare la parola a nessun altro esponente di tale Gruppo a meno che non fosse in dissenso, come sta avvenendo

Sono parole che avrei voluto sentire, che ho sollecitato anche ieri con le votazioni di altri emendamenti che erano sempre su questo tema, su questo passaggio che si ripete perché la legge

politica e civile che ha ispirato la senatrice Soliani a fare quell'intervento e a dire quelle parole poc'anzi. Era doveroso, era importante che ci fosse questo passaggio. Mi aspetterei lo stesso passaggio - visto che gli emendamenti sono stati diversi - da tutte le altre componenti della maggioranza attuale. Vorrei che tutte le altre componenti della maggioranza e del Governo maggioranza e del Governo - che condividono l'esperienza governativa, in questo momento con la senatrice Soliani, che condividono i principi ispiratori del programma e adesso, in questa situazione

l'emendamento non venga accettato. Nei motivi ispiratori però e nel ragionamento che porta a dire "no" certamente ci sarebbe una spaccatura forte, frontale, diretta e chiara nella maggioranza. Ciò che non posso condividere - e ciò che potrebbe essere un arricchimento al dibattito - sono le motivazioni con cui la senatrice Soliani arriva al suo «no» a questo emendamento come agli altri emendamenti: viene citata la Costituzione. Certo, la parità è garantita in Costituzione, in Costituzione, ma la Costituzione non parla degli studenti, la Costituzione parla dei cittadini. I soggetti della scuola non sono solo gli studenti; sono gli studenti, le famiglie, gli insegnanti, le forze sociali che concorrono alla scuola,

è un dato di fatto. Va bene, ma la scuola o la Costituzione non può essere trascinata o tirata per la giacca solo da una parte.

e non ci sarebbe il problema probabilmente se la parolina "paritaria" fosse inserita nel documento. Se invece c'è questo accanimento, se c'è questa situazione è probabilmente perché il problema c'è. Poi, possiamo nasconderci dietro il dito nel dire: «No, non c'è. Sì, c'è». Alla fine, però, vuol dire che il problema c'è.

a sostenere l'esame presso le scuole statali, erano componenti della commissione d'esame. Quindi, se vale per uno, non si capisce perché non debba valere per tutti gli altri.

a giudicare gli studenti delle scuole statali o viceversa gli insegnanti delle scuole statali vanno a giudicare gli studenti delle scuole paritarie, a parte che questa seconda ipotesi c'è da sempre.

non è che non ci interessi; fa parte del sistema, ma non risponde ai princìpi, ai meccanismi dell'altra tipologia, perché per definizione è privata, viaggia su canali propri, vive per conto proprio, ha regole

in un'altra, pubblica o privata. Non è se la stessa cosa che chi insegna in una scuola privata abbia perciò solo i titoli che possono essere vantati da chi insegna in una scuola pubblica,

i fideisti non hanno mai paura di sbagliare, seguono la stella filante e finché fila la stella filano anche loro. Non sono della stessa opinione e mi permetto qualche volta di non avere le stesse opinioni del mio Gruppo, che è così liberale che consente, a chi non è d'accordo su temi che investono la coscienza, di esprimersi liberamente e di fare con questo il proprio dovere parlamentare. Il parlamentare, infatti, rappresenta la Nazione senza vincolo di mandato. Non è, onorevoli conformisti, che si sta d'accordo per fare finta di tirare quattro paghe per il lesso della maggioranza.

Signor Presidente, poiché ritengo che il tema sia fondamentale non sono intervenuto in dissenso tecnico, dato che in quest'Aula anche un voto è prezioso. Mi auguro che qualche collega rifletta sull'importanza di questo voto e magari, anche se non cambia idea, almeno ascolti le mie considerazioni. *(Applausi dal* situazione costituzionale nel sistema scolastico è diversa da quella alla quale si modellano degli stereotipi del passato: scuola privata e scuola pubblica o statale. La legge di parità scolastica ha segnato un traguardo e un punto di partenza nuovo rispetto al passato, perché ha riconosciuto alle scuole paritarie le stesse funzioni e la stessa dignità delle scuole statali e ha creato, quindi, un sistema pubblico unitario accanto a quello che rimane, e non potrebbe essere certamente cancellato, un sistema scolastico privato che segue altre strade, altre vicende, altre verifiche che non sono in gioco negli emendamenti presentati su questo provvedimento. Allora, se così è, si è al di là del dettato costituzionale, che comunque prevede la possibilità di un regime di parità, imponendo però alle scuole paritarie di rispettare la dignità scolastica dell'alunno

Tra questi, vi è il riconoscimento dell'assoluta equivalenza tra l'organizzazione della scuola statale e quella della scuola paritaria, cioè di tutti i soggetti che operano nel sistema scolastico pubblico. Se non lo si comprende si può anche fare riferimento a situazioni che nulla hanno a che vedere con le problematiche di cui oggi discutiamo

Vi è solo una chiara ed esclusiva ragione politica, nell'ambito della maggioranza di centro-sinistra, perché alcune forze appartenenti alla sinistra radicale non vogliono sentir parlare di scuola paritaria. Questa è la realtà di scelte così negative. Ebbene, se così è, desidero fare un appello a chi non appartiene alla sinistra radicale, comunista o postcomunista, e a quella radicale ecologica.

testo. È noto a tutti che questa maggioranza vuole escludere dai commissari esterni i professori abilitati che insegnano nelle scuole paritarie, mentre mentre gli insegnanti di scuole statali, anche soltanto in qualità di supplenti temporanei non abilitati, possono partecipare come commissari esterni agli esami di Stato. Siamo veramente alla pazzia

Presidente, colleghi, ancora una volta, si assiste ad un accanimento non terapeutico ma, a mio avviso, schizofrenico della maggioranza e del Governo contro quelle categorie

si possono annidare simpatizzanti del centro-destra, hanno riportato una vittoria sul Giano bifronte Rutelli, che all'inizio sulla tassa di soggiorno disse «I soliti piagnistei, va bene»" e invece ieri sera, in televisione, con una faccia tosta allucinante,

Per Rutelli ce ne saranno tante nel corso degli anni: basta vedere i miliardi che ha dispensato ad un cinema che al massimo può accogliere mille spettatori, mentre dimentica altri tipi di cinema.

docenti anche precari, purché provenienti dal settore statale? Ci sembra l'ennesima ingiustizia contro quella scuola alla quale noi, sin da oggi, faremo sentire il distacco e l'odio che la maggioranza ed il Governo mostra nei

dell'assurdo legislativo, dell'irrazionale; non c'è neanche bisogno di tirare fuori la Costituzione, in questi casi: basta il diritto dei lavoratori, basta

assunto chi è a tempo indeterminato e non chi è a tempo determinato, quando poi magari l'esperienza, le storie, la professionalità sono le medesime. Mi permetto di fare

Non è un riconoscimento, ma una concessione e bene fa lo Stato, perché le scuole paritarie devono attenersi a quei princìpi, perché la parità è un diritto e contemporaneamente un dovere. Questa la mia precisazione.

Presidente, penso che il confronto ed il dibattito che si stanno sviluppando in quest'Aula su questi temi siano esplicativi della serietà

con un intervento (nelle mie parole non c'è nessun intento di offesa nei suoi confronti)

questi temi. Vorrei richiamare anche l'attenzione di altri colleghi, come il presidente Fisichella, che pure è stato un cultore

hanno riscontrato la sua attenzione anche nell'ultima sua fatica saggistica. Ebbene, senatrice Soliani, la scuola cosiddetta privata, che poi in realtà privata non è in questo Paese, ha avuto grandi tradizioni. Basti ricordare quello che è stato il significato delle scuole non statali, salesiane, per quanto riguarda gli istituti professionali, che hanno contribuito enormemente al processo di industrializzazione di questo Paese e che costituivano un sapere tecnico collettivo di grande rilievo. Mi voglio soffermare anche sulla tradizione cattolica, popolare, dell'Opera dei Congressi, sulla tradizione culturale, di valorizzazione dei corpi intermedi

rinnegata dalla componente cattolica della sinistra. È inutile poi venire in Aula a rivendicare la legge n. 62 del 2000.

Fu la nostra opposizione a mitigare i contenuti di quella legge che doveva essere punitiva verso la scuola non statale. Grazie. a concetti, a culture punitive e, come ho detto anche in un precedente intervento, neogiacobine. Ecco, allora, di cosa stiamo discutendo ed ecco perché in quest'Aula, all'improvviso, si è infiammata la discussione.

quindi non hanno l'abilitazione professionale a insegnare, certificata dallo Stato. Tuttavia, pur essendo privi della certificazione dello Stato sulla loro professionalità, possono, soltanto perché hanno ottenuto una supplenza in una scuola statale, entrare a fare parte delle commissioni di esame. C'entrano poco la scuola parificata o paritaria e la scuola statale: qui è in gioco una discriminante per i cittadini di questa Repubblica. Chi è abilitato e insegna in una scuola paritaria non può far parte delle commissioni delle scuole statali. La discriminante colpisce dunque un cittadino di questa Repubblica che è in possesso del titolo statale ma, per il semplice fatto che si trova a operare in una condizione diversa di lavoro, viene discriminato. In questo sta la gravità. È inutile che la relatrice

di sensibilizzare l'intera opinione pubblica, non solo quella cattolica, su queste vostre politiche discriminanti, su queste vostre politiche neorazziali. Qui sta il nocciolo duro del discorso che stiamo affrontando in quest'Aula.

intervento della relatrice. Dico questo perché credo che quando si discute di questi temi non vi sia nessuna disputa confessionale in gioco. Il tema in discussione non è l'appartenenza religiosa di chi si iscrive a scuole non statali o di chi insegna in queste scuole, ma è, in ultima analisi, la libertà di educazione, che è un valore laico, non confessionale e, in quanto tale, non può non essere condiviso da chiunque. Non sono in gioco stelle filanti, come è stato detto, da seguire anche perché altra tipologia di stella veniva seguita, non certamente quella filante. Si tratta di riconoscere pari dignità a qualsiasi tipo di offerta di istruzione, anche quella non statale, che non coincide con quella confessionale cattolica (anche se quest'ultima ne costituisce una larga parte), non coincide con istituti cattolici (che pure sono preferiti da ampi strati di popolazione non credente). Esiste un'offerta formativa non statale che fa riferimento ad altre confessioni religiose, ma anche ad offerte formative non confessionali, che pure hanno una qualifica non statale. La libertà di educazione chiama in causa, in definitiva, la titolarità dell'educazione, che non può non collegarsi con il diritto da riconoscere ai genitori e non con un potere da riconoscere allo Stato. Questi sono i temi in discussione, rispetto ai quali - lo ripeto con il massimo equilibrio - non comprendo un risentimento come quello dimostrato dalla relatrice, che mi pare eccessivo, perché su questo, come su altri temi, l'ala cosiddetta moderata del centro-sinistra vota e, alla fine, manifesta nei fatti concordanza di opinioni con la parte più radicale della sinistra. Ciò è accaduto quando si discuteva, nonostante tante proclamazioni iniziali, del finanziamento alla ricerca sulle cellule staminali ricavate dagli embrioni e, alla stessa maniera, accade ora che si discute dell'innalzamento della soglia che segna il confine tra l'illecito amministrativo e l'illecito penale per la detenzione di sostanze stupefacenti. Il massimo che mi pare sia consentito a questa componente del centro-sinistra è manifestare un distacco iniziale soltanto verbale, salvo poi rientrare nei ranghi quando viene chiesto il voto. Certo, può provocare lo comprendo - che questa incoerenza venga sottolineata. Mi permetto di aggiungere, però, che ricordarlo e sottolineare questa incoerenza nei fatti è un diritto; non ammetterlo, magari con toni risentiti come quelli che abbiamo ascoltato, può essere una furbizia ma, per l'appunto, è una furbizia, non un atto di intelligenza.

credo che il collega Ranieri abbia ragione sul fatto che il tema è superato. Credo tuttavia che l'intervento del senatore Mantovano non possa

non esistano ragioni di principio che ostino al fatto che nelle commissioni d'esame di Stato possano esserci insegnanti abilitati delle scuole paritarie. Credo che se impostassimo la questione in chiave di principio non andremmo molto lontano. Ha ragione la senatrice Soliani quando dice che lo Stato ha il diritto-dovere di essere garante della competenza e della professionalità delle commissioni d'esame. Tuttavia, ha ragione chi nell'opposizione sottolinea come questa garanzia è data, innanzitutto, dal fatto che lo Stato ha abilitato quei docenti ad insegnare.

lo Stato, nella certificazione del livello di preparazione che hanno raggiunto gli studenti, è maggiormente garantito dal rapporto gerarchico e funzionale che si stabilisce con i propri funzionari e, quindi, con coloro che hanno con lo Stato un rapporto di dipendenza. Credo si possa discutere, trattandosi appunto di una questione di opportunità e non di principio, con pacatezza e - se mi si consente l'espressione - con laicità su questo tema.

il problema della scuola italiana non è principalmente questo. Lo voglio dire ai colleghi dell'opposizione e, in una certa misura anche ad una parte dei colleghi della maggioranza. Il problema della scuola italiana non è il rapporto tra scuola statale e scuola paritaria ed è impressionante come in tutte le sedi politiche e in sede parlamentare sembri invece che questa sia la questione centrale della scuola italiana. Abbiamo ben altri problemi e faremmo bene ad occuparcene assieme.

è fuor di dubbio che l'emendamento 1.183 comporti un costo aggiuntivo ma o avanziamo un'ipotesi di esami seri oppure rimaniamo come siamo, e mi spiego. Attualmente le commissioni sono tutte interne;

ASCIUTTI). Capite bene che questa vicinanza crea problemi significativi. La gran parte del Paese è formata da piccoli Comuni, dove al massimo ci

quella di spendere quattro soldi in più e creare problemi di campanile, oppure quella di tornare a una serietà nel Paese, se veramente ci crediamo? Se invece pensiamo di lasciare il sistema così com'è, tanto vale bocciare questo disegno di legge, che non serve ad un bel niente. Serve solamente a questo Parlamento e a questo Governo per dire che è stato fatto qualcosa per la scuola, per mandare un segnale al Paese. Ma quale segnale mandiamo?

infatti, totalmente divisi, tant'è che questo Governo, alla barba vostra, signori della maggioranza, con il cacciavite, come dicono Prodi e Fioroni, andrà a smontare la riforma Moratti attraverso circolari. Avremo una riforma fatta di circolari, che non passerà per il Parlamento. Che riforma sarà? Non lo sappiamo, nell'incertezza totale dei nostri studenti, delle famiglie e del Paese. Per questo motivo, signor Presidente, il voto di Forza Italia è favorevole.

su un punto che a me sembra di particolare rilievo. Nella scorsa legislatura e in quella immediatamente precedente abbiamo dedicato moltissime energie alla modifica del Regolamento,

Alla fine, con decisione unanime, abbiamo convenuto di dichiarare quell'emendamento improcedibile, a meno che senatori, segnalandosi attraverso la richiesta in questo senso con il sistema elettronico, non lo rendano procedibile, richiedendo esplicitamente che così avvenga. avvenga. A mio giudizio, signor Presidente, mi permetto di farlo notare, ciò significa che il Senato con il suo Regolamento ha voluto rendere chiaro che,

impegna il Governo a rinvenire adeguate risorse finanziarie per permettere, in futuro, di ricorrere a commissari esterni oltre i limiti previsti dal disegno di legge n. 960. L'ordine del giorno, votato all'unanimità, e, tra l'altro, firmato anche da alcuni componenti della maggioranza, testimonia chiaramente l'inadeguatezza della previsione contenuta nel presente disegno di legge e l'opportunità di questi emendamenti. L'ordine del giorno dice esattamente quello che anche noi affermiamo.

collusioni o inimicizie a danno degli allievi di una determinata scuola. Faccio un esempio molto concreto: è evidente che, laddove vi siano due licei che insistono sulla stessa area, ci potrebbe essere essere un interesse dei commissari esterni a far vedere che la preparazione di quegli studenti è inadeguata affinché le famiglie iscrivano i ragazzi al proprio liceo; oppure ci possono essere accordi e intese per una sorta di solidarietà ambientale, sapendo che l'anno successivo può toccare al collega essere in commissione nella propria scuola.

La novità è che inserisce nell'ambito regionale e interregionale la la distribuzione o l'assunzione dei commissari che giudicano i ragazzi negli esami di Stato.

non siamo di fronte a un esame serio, ma a un provvedimento tampone. Lo abbiamo condiviso in queste settimane; siamo realisticamente convinti che questa discussione sia inutile per adesso, ma

era il minimo dei compensi per i commissari interni delle scuole, anzi soprattutto per i presidenti che venivano mandati in una commissione che era composta

ad un'impostazione seria, cioè ad un esame finale che è uno strumento di giudizio, di valutazione di competenze, di professionalità e di livelli culturali,

che questa maggioranza ha stabilito per la finanziaria: una logica di taglio, soprattutto nel mondo della scuola. Vi sono logiche di taglio anche in quell'invito a non bocciare più per risparmiare qualche decina di milioni di euro in più. Da una parte, quindi, la maggioranza chiede che venga risparmiata qualche decina di milioni di euro in più per promuovere anche i somari e, dall'altra parte, siamo di fronte ad una riforma dell'esame di Stato - che nessun ha chiesto, che nessun vuole e che tutti riteniamo inutile, se non per sciacquarci la bocca, per lustrarci gli occhi di fronte al mondo della scuola e per dire che si è fatto qualcosa - che ci costerà 100 milioni di euro in più. Non condividiamo quella logica, ma non perché non la si condivide, perché le parole del senatore Asciutti hanno ben inserito il senso del suo provvedimento e quindi il nostro voto di fronte a questa situazione non può che essere negativo.

respinto, che riguardava la possibilità che i commissari esterni si potessero muovere nell'ambito nazionale, viene incontro a quanto il senatore Davico

d'esame: quelli del Nord rimarrebbero al Nord, quelli del Sud rimarrebbero al Sud. È un modo di venire incontro alle esigenze che ha espresso or ora, a nome della Lega, il senatore Davico.

del livello di promozione educativa all'interno di una società. In quest'Aula, nessuno potrà negare che la Francia sia un Paese profondamente laico,

ad un tipo di scelta educativa competitiva e liberale - ma anche in quella che fu la patria dello statalismo. La senatrice Soliani altri colleghi della maggioranza penso che lo abbiano capito, tant'è vero che hanno ritenuto di intervenire nel presente dibattito per tentare di attenuare le responsabilità derivanti

della serietà del confronto politico che si sta sviluppando in Aula. Accade sempre così: nelle fasi di transizione storica e politica, i contemporanei, in genere, non avvertono i profondi mutamenti che avvengono nella società e li vivono come semplice cronaca. Questa fa parte, appunto, di quella che potremmo definire l'inconsapevolezza diffusa, in una fase storica come questa, che è presente in tutti gli schieramenti politici: è inutile negarlo. Allora, l'opzione della scelta formativa, che è collegata al livello di competitività, provoca una crescita del sapere collettivo all'interno di una società e di un Paese. Il motivo per cui la scuola italiana è regredita al livello dei Paesi più arretrati del Sud America è proprio questo, perché non essendovi competitività tra scuola non statale e statale

ragioni, è inutile nascondersi dietro il dito degli sciocchi, facendo credere che stiamo discutendo, cari senatori dell'opposizione, dell'assegno che

questa scuola iperstatalista ha portato il Paese a non essere competitivo come sistema nei confronti delle economie dei Paesi avanzati. La verità è che non siamo competitivi non solo, come

riferiscono alla Presidenza ed indicano eventuali anomalie nell'esercizio del voto. Quindi, la prego di astenersi perché la Presidenza governa questa Aula secondo il Regolamento. Invito

chiusa la votazione.

paritarie e scuole statali che fanno parte integrante del servizio scolastico pubblico nazionale; poi, si avranno le scuole esclusivamente private ma non più legalmente riconosciute.

istituzioni scolastiche e non scolastiche, esterne alle istituzioni, il mondo della scuola, il mondo delle agenzie formative. Sono convinto e siamo convinti che

della valutazione corretta, giusta del termine del ciclo degli studi passi, o debba passare, attraverso un atto di coraggio, che è l'abolizione del valore legale del titolo di studio.

un percorso, un'operazione istituzionale e legislativa più complessa.

Pregherei i colleghi di sedersi e di abbassare il tono della voce, perché ha ragione il collega senatore che parla: è difficile parlare ad un'Aula con questo livello di brusìo. Grazie. DAVICO *(LNP)*. La ringrazio, signor Presidente. Siamo sicuri, mi domando, cercando di fare questo breve ragionamento, che una persona, un ragazzo, un nostro cittadino

da un unico esame finale? Siamo sicuri che con quell'esame gli venga rilasciato un titolo che lo giudica, che lo valuta completamente? Le strade che le scuole hanno scelto ormai sono altre, indipendentemente dal nostro dal nostro giudizio e dalla nostra legislazione. La strada principale è quella della certificazione: le scuole hanno superato il valore legale del titolo di studio con la certificazione. Le università hanno superato il valore legale del titolo di studio con i test di accesso. Il mondo del lavoro ha superato il valore legale del titolo di studio con sistemi di di vario genere, con cui si assumono le persone, ma la cui formazione comunque continua o viene approfondita o viene recuperata. Il mondo delle professioni ha superato il valore legale del titolo di studio con il praticantato, con esami di accesso alla professione.

Quindi, ci sono prove di valutazione del percorso al quarto anno scolastico oppure altre prove per l'accesso all'università al quinto anno. Ecco, ci vorrebbe un atto di coraggio in questo senso; ormai tutti sappiamo che quel titolo, quel pezzo di carta, quel timbro non ha più il valore che poteva avere quando il nostro Paese stava costruendo il proprio sviluppo dal dopoguerra in poi. Quindi, di fatto il valore legale del titolo di studio è superato. Il superamento vero, anche legislativo, del valore legale del titolo di studio, porterebbe all'autonomia piena, perché a quel punto non sarebbe più il pezzo di carta

la certificazione delle competenze, del livello culturale, professionale, di maturità che si è raggiunto, ma questo presuppone una revisione di tutto il sistema scolastico. Se n'è parlato in quest'Aula, in occasione di questo articolato dibattito, ma ci sarebbe bisogno di un'impostazione, di una riforma complessa del mondo della scuola, soprattutto della scuola superiore, in questo caso. A quel punto, la certificazione dei livelli raggiunti, il titolo di studio potrebbe avere un valore formale, comunque

la si sta costruendo, è importante lasciare la traccia. Si poteva anche ritirare questo emendamento (come tanti altri), però è importante lasciare la traccia, perché il futuro il futuro delle nostre istituzioni scolastiche, la garanzia della loro serietà, la vera autonomia, la certificazione vera di ciò che una persona, un ragazzo, uno studente è al termine di quegli anni di formazione e di impegno, penso veramente che possano passare attraverso un cambiamento vero, un cambiamento grande. è uno dei punti: non più lo Stato che dà il pezzo di carta ma un qualcos'altro, quindi questo emendamento rappresenta un segnale della volontà della richiesta di un passaggio. veramente i colleghi di rispettare la tradizione del Senato. Tendenzialmente i colleghi senatori devono stare seduti e possibilmente non dare le spalle alla Presidenza, anche perché credo che l'istituzione Senato sia una cosa importante per tutti e non riguardi le parti. Cerchiamo di dare un decoro alla nostra Aula e ai nostri lavori, rispettando almeno un minimo di tradizione di questa straordinaria assise. Grazie, colleghi. Presidente, la ringrazio. Mi piacerebbe, nell'ambito della dichiarazione di voto su questo emendamento, sentire il parere dei colleghi, dei Gruppi, perché penso sia il il riferimento nuovo che dovrà essere studiato, valutato e proposto, per superare quei problemi strutturali, storici, di cui abbiamo parlato nell'ambito di questa discussione.

il valore legale dei titoli di studio, questione che dispone - com'è noto - di una vastissima letteratura. trovo qualche difficoltà a conciliare la prima parte di questo emendamento con la seconda. Mentre, infatti, nella prima si dice che il titolo certifica il possesso delle competenze didattiche, nella seconda parte si dice esattamente l'opposto, cioè che ha valore esclusivamente formale. Se il titolo certifica il possesso delle competenze didattiche, esso ha valore sostanziale, non formale. Credo pertanto che l'emendamento non si possa accogliere.

Prendendo visione dell'elenco dei senatori non partecipanti alla votazione con procedimento elettronico n. 9, ho potuto notare il mio nome. Comunico alla Presidenza che sono stato in Aula dalle ore 9,30 di questa mattina fino adesso senza mai uscire e partecipando a tutte le votazioni.

anche perché provengo da una città come Napoli che ha conosciuto, conosce e vive, nella sua complessità, la storia e la tradizione

una tradizione, in un certo senso, meno iperliberista e liberale verso questo tipo di impostazione del problema. Vorrei, tuttavia, ricordare

attuare, come processo innovativo, proprio una rottura con il passato perché, sostanzialmente, sosteneva un percorso formativo non solo certificato, ma vissuto dall'istituzione scolastica in tutte le fasi della vita dello studente. Il percorso formativo, cioè, veniva attuato e vissuto con la presenza, la partecipazione non solo del corpo docente ma anche delle famiglie.

sulla necessità di una diversa lettura di quanto è avvenuto nella precedente legislatura. Non riesco a capire perché proprio la Lega, che ha votato e condiviso quel tipo di impostazione in contrasto con l'attuale maggioranza di Governo, ora debba rinnegare quanto di buono è stato fatto e attuato dal Governo Berlusconi. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo dell'UDC, anche se riteniamo che questa interessante provocazione che il senatore Davico ci pone questa mattina e che ha già posto in sede di Commissione possa diventare argomento di una riflessione ben più vasta, ha già toccato le Commissioni e le Aule del Parlamento. Certamente dovremo rivedere completamente l'impianto del nostro sistema formativo per arrivare ad altre conclusioni: questa certificazione, che comunque lo stesso emendamento richiama, sia cioè fatta a sbarramento del processo formativo prima dell'accesso alla professione, come avviene in molti Paesi del mondo. Certamente, con l'attuale sistema, saremmo assolutamente impreparati nell'accogliere un emendamento di questo tipo.

certamente non è un problema banale, ma centrale della discussione sul futuro del nostro sistema formativo. Alleanza Nazionale ritiene che, per quanto riguarda il sistema universitario, certamente si possa andare verso una progressiva abolizione del valore legale, magari con un'autonomia sempre più rafforzata delle università. Per quanto riguarda il sistema di

determinano l'aggregazione del nostro popolo attorno ad una identità. Voglio soltanto fare un esempio molto concreto: si potrebbe arrivare al paradosso che chi riveste ruoli

credo che un passaggio di questo tipo, sopratutto in questa fase storica, correrebbe il rischio di indebolire l'unitarietà del nostro Paese. Pertanto, Alleanza Nazionale voterà contro questo emendamento.

Signor Presidente, colleghi, avevamo proposto una serie di emendamenti per migliorare l'articolo 1, che sono stati respinti nella foga della maggioranza di portare a casa con urgenza un provvedimento che non condividiamo nei suoi presupposti fondamentali.

dei giovani che attendessero di conoscere quali provvedimenti questo ramo del Parlamento intenda assumere a vantaggio della propria formazione, credo che il loro giudizio

è difficile parlare con tanto brusìo. Dicevo che questi giovani si trovano davanti a un Parlamento che discute di rigore senza aver preventivamente discusso di opportunità, senza aver preventivamente discusso di ciò che obiettivamente serve per renderli competitivi. Vedete, assistiamo ad un mutamento delle esigenze del nostro Paese in rapporto alla globalizzazione della crescita. crescita. Prima la concorrenza e la competizione erano all'interno dei Paesi, ora sono all'interno dell'Europa. I nostri giovani competono con quelli delle altre Nazioni europee e quando tale competizione non può avvenire ad armi pari, quando gli strumenti a disposizione dei nostri giovani non sono gli stessi di quelli messi a disposizione dei giovani degli altri Paesi europei, tale competizione diventa falsa e la classe dirigente del nostro Paese non può concorrere con quella degli altri Paesi nella costruzione della classe dirigente europea.

Abbiamo registrato in questi due giorni di dibattito la costante presenza in Aula del Ministro Guardasigilli di uno dei sette Paesi più industrializzati del mondo. Sembra quasi che il ministro Mastella non abbia da pensare allo sciopero in corso degli avvocati quasi che non avesse grandissimi problemi che riguardano proprio il mondo della giustizia. Siamo stati onorati anche della presenza del Ministro della sanità, la quale, tra una telefonata e l'altra, avrà provveduto alla nuova decretazione relativa

deve portare a casa tale provvedimenti così com'è, senza la possibilità di emendamenti da parte dell'opposizione. Questo, infatti, non è un provvedimento amministrativo,

di mera ideologia. Non ha importanza se i colleghi della maggioranza hanno una diversa visione del mondo della scuola, perché diversa è la visione

le posizioni dell'intimo pensiero, le posizioni di coerenza che dovrebbero caratterizzare ciascuno di noi. *(Applausi dei senatori avere due sfere morali: la sfera personale e quella pubblica. Lo dico con affetto agli amici centristi della maggioranza di centro-sinistra: fino a quando potrete continuare ad avere il doppio binario della vostra coscienza? Leggiamo sui giornali che siete coerentemente contro l'utilizzo della droga e siete, poi, incoerentemente presenti in Aula a votare qualsiasi provvedimento vi venga proposto. Non è possibile che nella sfera privata e nel vostro dialogo con il mondo cattolico dichiarate che siete per una scuola paritaria, che siete per una scuola delle opportunità, che siete per una scuola che riconosca la centralità del discente e quindi dell'uomo nel sistema formativo e poi venite in Aula e vendete il vostro voto e il vostro consenso sull'altare della strategia politica, della compattezza della maggioranza! Non fate ancora mercimonio del vostro pensiero! Non fate ancora mercimonio di ciò che dovreste testimoniare anche con il voto in Aula!

nella notte nera in cui tutte le vacche sono nere, non si fa l'interesse del Paese, non si può tirare avanti. Non si può soltanto tirare avanti, in in modo che il Governo Prodi resista. Nell'attesa che il Governo Prodi sopravviva, non possiamo realizzare guasti così profondi per il Paese.

Lo Stato veramente laico e non confessionale è quello che garantisce ai propri giovani la formazione scolastica, la competitività, la realizzazione del proprio io attraverso lo strumento della scuola. Allo Stato laico Allo Stato laico non interessa se concorrono alla formazione del giovane le strutture pubbliche o quelle private: allo Stato laico interessa che per quel giovane vi sia la migliore formazione possibile. È per questo che oggi siamo costretti a votare contro l'articolo 1 e ad opporci a questo provvedimento.

Grazie.

Le motivazioni sono semplici: l'articolo 2 prevede una «delega» al Governo «in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione dei risultati di eccellenza». Non avremmo niente in contrario se fosse cassata la lettera *c)*, perché tale lettera parla di «valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari». Questo è grave, perché lede in maniera forte l'autonomia universitaria, in quanto si delega alle prove dell'esame di Stato la possibilità per gli studenti di partecipare a un corso di laurea dove è prescritto un concorso di ammissione.

che hanno raggiunto il massimo livello di istruzione. Se questi studenti dovessero poter partecipare, senza concorso o con un peso significativo,

sono studenti provenienti dal liceo classico, dal liceo scientifico, dagli istituti industriali e dagli istituti professionali. Come si fa a distinguere il 100 su 100 di un corso rispetto ad un altro? È solo l'autonomia universitaria che può decidere, con un esame, quali

la legge delega. Certo, se questa maggioranza oggi prevede che dodici mesi siano già troppi perché il

realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica

le parole «definendo altresì, in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico‑scientifiche». Chiedo di cassare questo periodo, perché mi chiedo: come si fa in legge a dire che vanno valorizzate esclusivamente le discipline tecnico-scientifiche, come se questo Paese avesse all'improvviso dimenticato la sua storia? Questo Paese ha una storia, assieme a quella francese, dove sono stati nel tempo privilegiati il percorso e gli studi classici. Oggi si vuole realizzare un'inversione di tendenza. Ma perché metterlo in legge? Questo è un assurdo. È un emendamento che chiaramente viene da una parte della maggioranza, dove Governo probabilmente ha dovuto subire, ma veramente è un assurdo in termini, come se la nostra cultura dovesse essere indirizzata esclusivamente alle materie scientifiche.

il senatore Fluttero, pur essendo sempre in Aula e votando regolarmente, risulta costantemente assente. Allora, vorrei pregarla di chiamare i tecnici e - se è possibile - di rimediare immediatamente, altrimenti sospendere i lavori.

risulta assente. Credo che questo valga per noi, ma anche per voi della maggioranza. Non vedo perché si debba far polemiche anche per queste cose.

Non è che quando si è in maggioranza il voto vale doppio! Senatrice Serafini, le spiace togliere la tessera al suo fianco?

Prendiamo atto del fatto che lei intende ripetere questa controprova, ma quello che sta accadendo è un po' grave. Sono sempre rispettoso dei controlli reciproci, ma o ci diamo regole - che vi sono sempre state - o saremo costretti a mutare il nostro atteggiamento in Aula.

questo è un fatto incontestabile, sempre acclarato e realizzato in tanti anni di attività del Senato. È la prima volta, nella presente legislatura, che assistiamo a certi atteggiamenti, come quelli ai quali abbiamo assistito poc'anzi, da parte di parlamentari che lasciano i propri banchi

perché ove si dovesse realizzare un ulteriore episodio come quello che è testé accaduto alle mie spalle, saremo i primi ad occupare i banchi della maggioranza. Senatore Schifani, proprio prima del suo intervento la Presidenza aveva richiamato la senatrice Donati a recuperare il proprio posto.

Spesso queste passeggiate negli emicicli ‑ forse capita più alla Camera, dove vi è maggior istintività giovanile ‑ si concludono con scazzottate, che credo sia assolutamente sconveniente sollecitare.

Senatore Garraffa, anche quando non si sta votando deve farci sentire le sue capacità da tenore? VALDITARA *(AN)*. Ritengo che la norma di cui proponiamo l'abrogazione, o comunque una riformulazione, sia gravemente lesiva dell'autonomia del sistema universitario, perché prevede sostanzialmente che la votazione conclusiva della maturità dia un punteggio ai fini dell'ammissione all'università. Un meccanismo di questo tipo, fra l'altro, non distingue fra i vari tipi di scuola

all'indebolimento di quei meccanismi selettivi che le università da tempo hanno avviato e, dall'altro, a incoraggiare soprattutto in determinati ambiti, votazioni particolarmente elevate per garantire, magari a scapito di altre realtà,

Purtroppo non abbiamo approvato alcuni emendamenti che avrebbero consentito una maturità più trasparente, più oggettiva e più omogenea su tutto il territorio nazionale ( penso in particolare a quelli relativi alla terza prova). Ora, di fronte ad una maturità che non è in grado - a mio avviso - di determinare una adeguata selezione credo che danneggeremmo il percorso universitario e rischieremmo di penalizzare quegli studenti che studiano nelle scuole più serie e meritocratiche,

del godimento di alcune facilitazioni relative per esempio al diritto allo studio, alle residenze universitarie e a quant'altro, che in questo caso credo possano sicuramente ammettersi.

ancora uno spiraglio residuo di dialogo e di comprensione tra maggioranza ed opposizione su questo tema perché ciò darebbe comunque l'opportunità di prolungare la riflessione su questo disegno di legge, una riflessione che è sostanzialmente mancata. È vero che abbiamo dedicato molto tempo alla discussione in Aula, ma è anche vero che la discussione sugli emendamenti si è sempre iniziata con un elenco secco di no da parte della relatrice - praticamente su tutti da parte del Governo vi è stato un breve intervento per lo più dedicato ai ringraziamenti e molto poco ai contenuti e alla sostanza. anche che si vive un passaggio politico alla vigilia della finanziaria non certo favorevole ad un clima di dialogo, ma credo che questo argomento, come è stato detto molte volte, doveva uscire da una logica di pura contrapposizione per diventare un'occasione più distesa ed interessante per affrontare un argomento che supera la contingenza ad un anno e che ci si augura debba durare qualcosa di più dell'arco di una legislatura, come è stato invece per tutti provvedimenti che hanno riguardato le riforme degli esami di maturità negli ultimi anni. Non si può però non stigmatizzare in questo passaggio un comportamento incredibile da parte della maggioranza che ha bocciato anche i cosiddetti emendamenti «camomilla», quegli emendamenti che non avrebbero svegliato nessuno - e sicuramente non il clima di contrapposizione, che almeno come Gruppo UDC su questa legge non desideriamo - ma che sono stati tutti regolarmente respinti. Faccio riferimento ad alcuni emendamenti di natura puramente tecnica se non lessicale. Anche su quelli non vi è stata alcuna possibilità di dialogo. Vorrei poi sottolineare che i pochi emendamenti che sono stati presentati

non vi sia la benché minima volontà di comprensione. Cisaremmo aspettati invece che fosse la stessa maggioranza, con un briciolo di buonsenso, a dire che non era possibile applicare questa legge in corso di anno scolastico, portandola praticamente a ridosso delle vacanze di Natale quando si segna sostanzialmente la metà dell'anno. Se fosse stata approvata prima avrei potuto comprenderne il motivo, ma già adesso mi sembra fuori da ogni buon senso. La stessa relatrice, che secondo me ha mancato alcuni appuntamenti in questo dialogo, è invece intervenuta riguardo all'emendamento presentato dal sottoscritto e dal collega Buttiglione riguardo alla possibilità di utilizzare i docenti delle scuole paritarie nelle commissioni di esame anche delle scuole statali. Siamo particolarmente onorati per la comprensione e l'attenzione che la relatrice ha voluto dare nei confronti del nostro emendamento, ma non si può in nessun modo condividere l'intervento che ha fatto. Mi aspettavo, senatrice Soliani, che il suo intervento fosse finalmente di contenuto e di merito riguardo all'argomento in discussione e non invece una cortina fumogena sollevata su una questione di natura religiosa ed ideologica che non avevamo in alcun modo posto, ma che a questo punto siamo costretti a porre anche in sede di dichiarazione di voto. È stato portato come esclusivo argomento

nei confronti del nome di Dio. Io mi sento, signor Presidente, di difendere per lo meno la posizione dei colleghi del mio Gruppo, perché sicuramente da parte dei colleghi del Gruppo dell'UDC non c'è nessuna strumentalizzazione del nome di Dio. Se le terminologie in uso, quelle alle quali credo la senatrice Soliani facesse riferimento, sono i teocon, i teodem e i teopop, la senatrice dovrebbe guardarsi all'interno del suo Gruppo, in modo particolare all'interno del Gruppo della Margherita, relativamente all'utilizzo dei termini teodem e teopop, che voi avete coniato.